dopo aver vissuto intensamente l'esperienza cruciale del passaggio ordinamentale tra gli anni 1943-1948, ebbe la straordinaria capacità di leggere in profondità tutte le grandi ideologie di massa che hanno percorso la seconda parte del Novecento in Italia. La sua opera di storico va ben al di là dell'analisi del movimento cattolico e dei suoi sviluppi partitici e i numerosi contributi scientifici denotano una non comune versatilità nell'analisi della storia economica e sociale, dei processi evolutivi determinati dai movimenti politici e, in generale, dalle aggregazioni partitiche in epoca statutaria. La sua stessa vicenda personale, che lo vede prima combattere sul fronte africano ad El Alamein e poi entrare a far parte della Resistenza, contribuisce alla maturazione di una sensibilità e capacità di comprensione storica tanto dei singoli momenti di rottura degli equilibri, quanto dei lenti processi di cambiamento e di mutazione. Del resto, la sua carriera accademica, avviatasi col conseguimento della libera docenza in Storia contemporanea nel 1958, lo vedrà insegnare nelle università di Padova, di Salerno - di cui fu anche Rettore - e, quindi, di Roma. L'attenzione dello storico per l'evoluzione del Mezzogiorno d'Italia, si accompagna negli anni più produttivi delle sue ricerche alla pubblicazione di opere decisive che rappresentano, ancora oggi, un indefettibile punto di partenza per la comprensione del movimento cattolico in Italia. Ne sono evidente testimonianza prima la sua «Storia del Partito popolare italiano» del 1958 e quindi la successiva «Storia del movimento cattolico» del 1966. Dal 1979 ad oggi è stato Presidente e poi Presidente onorario dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma, in cui le sue iniziative scientifiche hanno trovato il naturale sbocco nell'approfondimento della funzione del Partito popolare in Italia: una forza politica capace di giocare un ruolo determinante nel processo di unificazione politica del Paese; un partito riformista ed inclusivo di larghe fasce della cittadinanza rimaste escluse dallo sviluppo economico differenziato per aree geografiche. La sua elezione a senatore avverrà soltanto nel 1987, ma egli sarà chiamato a contribuire in modo decisivo in un momento di passaggio delicato della vita della Repubblica. sarà proprio Gabriele De Rosa a ricoprire la carica di presidente del Gruppo parlamentare al Senato nei mesi dell'impervia transizione dalla Democrazia cristiana al Partito popolare italiano. Traspare così il legame indissolubile - sia nell'interpretare il pensiero religioso e politico di Don Luigi Sturzo, così come nel comprendere le cause della crisi dei partiti di massa nel nostro Paese tra la ferma consapevolezza delle peculiarità storiche che hanno contraddistinto il Sud dell'Italia e l'osservazione del decisivo tradursi nelle istituzioni repubblicane del pensiero cattolico. La ricostruzione del contesto economico e sociale è sempre volta a comprendere le direttrici dell'azione politica innovatrice che egli ha visto al servizio di un orizzonte politico di grande respiro. Ecco, allora, che le istituzioni diventano un cruciale punto di osservazione e dì studio nel tentativo di mantenere unito il tessuto civile di un Paese composto da molte anime e altrettante ideologie. Anche in questo non dobbiamo dilapidare la lezione dì metodo dello storico Gabriele De Rosa e cioè l'indagine sulla causalità storica, la quale, per quanto complessa e multiforme, non può mai cedere il passo a quelle letture di vago sapore antropologico che vedono nel cittadino italiano, e quindi anche nella politica italiana, un carattere irriducibile da cui discenderebbero vizi e virtù del nostro Paese. Onorevoli colleghi, la scomparsa di Gabriele De Rosa segna una perdita incolmabile per gli studi storici italiani e ci invita a ricordare l'esperienza di un uomo che, nella sua vita parlamentare, ha saputo tradurre costantemente il suo valore di studioso senza mai rinunciare a responsabilità e passione. passione. Invito, quindi, l'Aula ad osservare un minuto di silenzio.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare il Presidente

Con Gabriele De Rosa scompare non soltanto uno degli autorevoli membri di questa Assemblea, in più legislature, ma uno straordinario studioso del movimento cattolico, un acuto indagatore del vissuto religioso e della pietà; un testimone operoso dell'attualità e dell'impegno riformista dei cattolici italiani e della Democrazia cristiana. Sottolinearne l'opera con affetto e con gratitudine non è solo un dovere della cultura italiana, ma un impegno per quanti, riconoscendosi nel lavoro di ricostruzione del pensiero e del percorso storico dei cattolici italiani - cui egli ha dedicato il suo ingegno ed il suo impegno hanno tratto ispirazione e forza nelle difficili prove della politica.

con Gabriele De Rosa scompare una figura fondamentale di storico e di politico. È una sintesi della storiografia cattolica, ma un uomo di profonda onestà intellettuale e capace di aperture in senso pluralista. Abbiamo detto e ricordato che è stato parlamentare e si segnalò come uomo vicino al pensiero di don Luigi Sturzo e all'azione di Alcide De Gasperi. La sua voluminosa produzione gli ha permesso e ci ha permesso di scandagliare il rigore dello studioso e con la passione civile i più rilevanti fenomeni del nostro tempo. Attento osservatore e lucido indagatore dei movimenti che si sono succeduti nel secolo scorso, ha consegnato formidabili analisi e ha saputo sempre guardare alla storia con occhi accademici ma non freddi. Si è così meritato l'unanime apprezzamento di chi rifugge dalle ricostruzioni strumentali e piegate ai propri disegni. l'ultimo saluto al professor De Rosa, con lo spirito di chi sa che l'insegnamento, la comunicazione e il dibattito con i giovani sono stati al centro della sua esperienza e della sua esistenza.

poche parole per ricordare l'uomo, lo storico, il politico ma soprattutto il cattolico che ha testimoniato, nel corso della sua vita, un percorso lineare e trasparente. Non ho avuto una conoscenza profonda del senatore professor De Rosa, forse anche per motivi anagrafici, ma l'ho conosciuto come uomo mite e determinato; non è mai stato l'uomo per tutte le stagioni. Era molto vicino al Meridione

integerrime e pulite della prima parte della vita repubblicana con una seconda, i cui confini sembravano in quel momento avvolti da una nebbia consistente, nebbia che probabilmente egli non è riuscito a diradare neppure con i suoi studi preziosi.

che io voglio ricordare così come va ricordato: uomo libero

di servizio ma non al servizio delle bandiere. Insomma, un cattolico cui va il ringraziamento mio personale e dell'Italia dei Valori per quello che egli ha fatto

un intellettuale cattolico che ha profondamente segnato la ricerca e la cultura storica italiana ed europea, ma, insieme, un protagonista della vita civile e politica del nostro Paese. Sarebbe veramente difficile separare questi due aspetti. Tra le altre università, Gabriele De Rosa ha insegnato a Padova, nella mia università, ed i suoi studenti ricordano certamente il suo rigore nella ricerca storica, ma anche la passione civile la passione civile di una partecipazione politica che emergeva dalla sua presenza di studioso e di ricercatore. Sul piano della cultura storica ha avuto un grande merito, quello di aprire nel nostro Paese, fin dai primi anni

De Rosa: senza poter comprendere le radici culturali, sociali, organizzative e spirituali di un movimento che avrebbe costruito poi, con don Luigi Sturzo, il ritorno dei cattolici nella vita italiana dello Stato post-unitario insieme, l'eredità nella costruzione della vita democratica del Paese dopo il fascismo, il contributo dato alla formazione dello Stato democratico, la complessità di una storia politica italiana nel suo formarsi come giustapposizione di diversi filoni culturali - quello cattolico appunto, quello laico repubblicano e quello della sinistra marxista - complessità che ha saputo poi trovare le ragioni di un incontro nella costruzione delle nostre istituzioni democratiche, e alla cui costruzione il contributo di De Rosa non è stato secondario. Ma dell'importanza di De Rosa storico altri potranno dire in modo più autorevole; vorrei qui solo ricordare un lascito importante dell'opera culturale del professor De Rosa: lo sviluppo dell'istituto Luigi Sturzo, un istituto di ricerca e documentazione della storia del movimento cattolico che costituisce veramente un lascito di eccezionale importanza per le ricchezza delle fonti archivistiche che sono state lì Abbiamo detto dell'impegno di Gabriele De Rosa nella vita civile: ufficiale dei granatieri dell'Esercito italiano ad El Alamein; impegnato nella Resistenza contro il fascismo e, nell'immediato dopoguerra, nell'esperienza dei cristiani sociali; raccoglitore attento delle memorie di don Luigi Sturzo (in un bellissimo libro, "Sturzo mi disse", sono raccolti tanti pensieri di don Luigi Sturzo che sono di un'attualità straordinaria e che, grazie a De Rosa, ci sono stati trasmessi); impegnato poi nella Democrazia cristiana (intellettuale prestato, in questo caso, alla politica, come tante figure luminose dell'esperienza dei cattolici in politica, da Pietro Scoppola a Ruffilli, da Ardigò a Leopoldo Elia, che seppero tutti, usando gli strumenti di una piena laicità, portare con vigore nella vita pubblica idee e valori che si nutrivano dell'insegnamento cristiano, dell'esperienza del cattolicesimo sociale); per arrivare poi a questo estremo impegno di senatore, nel quale ebbe a svolgere, nel periodo più difficile e tormentato della storia politica recente del nostro Paese, il ruolo di Capogruppo della Democrazia Cristiana incarico non ricercato, ma assunto con generosità. Quindi, una lezione di grande attualità; nel momento in cui spesso nella cronaca quotidiana si tende ad asservire la ragioni della religione alle ragioni contingenti della politica, farebbe veramente bene a tutti noi rileggere le pagine così persuasive del professore senatore De Rosa su cosa vuol dire essere cattolici laici impegnati nella vita politica e culturale del Paese.

De Rosa, come il Presidente ha ben ricordato, entrò in quest'Aula nel 1987, al momento della chiamata a raccolta degli intellettuali d'area; io, che già lo conoscevo storiograficamente e come giovanissimo professore o aspirante professore di storia politica, lo ritrovai qui nel 1992).

giovanissimo e molto meno prestigioso capo del gruppetto dei senatori liberali, che all'epoca era un partito alleato con l'allora partito di maggioranza relativa) ricordo la straordinaria compostezza con cui il presidente De Rosa visse momenti terribili per tutti, ma in particolare per un uomo con le sue radici, la sua esperienza e la sua sensibilità. Rammento quando, insieme al capogruppo democristiano alla Camera dei deputati, l'onorevole Gerardo Bianco, De Rosa assunse l'iniziativa di scrivere molto importante nella quale si parlava di pentiti, di carcere, di visite ai pentiti nel carcere,

Credo che quel documento, purtroppo inevaso nella storia della Repubblica, sia ancora di una palpitante attualità

Luca. De Rosa, nato a Castellammare di Stabia nel 1917, nell'immediato dopoguerra militava nel Partito Comunista Italiano, scriveva su "Rinascita", aveva grandissima amicizia e sensibilità con uomini come Giulio Andreotti ed Andreotti ed Ossicini, un uomo che in questo palazzo se non in quest'Aula visse con intensità il dramma dell'autorizzazione a procedere nel caso di Andreotti. Qualcuno ha ricordato storiograficamente il contributo di De Rosa; vi sarà modo di tornare a ricordarlo, sottolineare che non lo limiterei alla storiografia politica in senso stretto. Penso che la grande storiografia debba molto agli studi antropologici di De Rosa sulla religiosità del Mezzogiorno d'Italia, ma anche nel Veneto, e che la grande storiografia sul movimento cattolico debba moltissimo al suo rapporto con Luigi Sturzo. Nondimeno, la preoccupazione espressa stamattina da Galasso circa una storiografia di De Rosa meno sensibile

e cortesia nei confronti di chi, come me - giovane che sedeva tra i banchi dell'estrema destra ed estremamente curioso - ogni tanto si avvicinava loro per chiedere e conoscere. Attraverso lui, ho conosciuto meglio don Sturzo e una storia del nostro Paese che oggi gli rende onore: era un uomo di grande trasparenza, onestà intellettuale

si deve, in parte, la povertà del nostro dibattito politico. Salutando in lui un grande maestro della nostra epoca e un grande maestro di democrazia, da cattolico convinto ricordo anche l'uomo che meglio ha fatto conoscere la storia del movimento cattolico e l'impegno dei cattolici in questo Parlamento. Il Governo si associa al cordoglio dei familiari. *(Generali ebbene, signor Sottosegretario,

Signor Presidente, sottosegretario Mantica, colleghi, in Sudan, Iraq, India, Nigeria, Indonesia, Pakistan, Cina, Egitto, Uganda, Congo, America Latina, Messico, Laos, Etiopia, Filippine e in altri Paesi, soprattutto islamici, le comunità cristiane vengono perseguitate: questo è quanto appare molto chiaramente dal Rapporto 2008 sulla libertà religiosa nel mondo,

impoverendo la sua sete di religiosità e cercando di mantenere le persone in uno stato di schiavitù. Nel nostro pianeta, la religione maggiormente discriminata e perseguitata è quella cristiana: nel mondo sono 2 miliardi i fedeli cristiani, 200 milioni dei quali vittime di persecuzione; possiamo stimare che tra il 75 e l'85 per cento degli atti contro una religione riguardi i cristiani. Questo quadro è desolante: le notizie di soprusi, violenze e persecuzioni si moltiplicano, disegnando una situazione dolorosa e antistorica, come se il tempo fosse tornato indietro di 2000 anni, all'epoca dell'impero romano. Le minoranze cristiane, quelle che vivono in terra di frontiera, anche se formate alla solidarietà, all'accoglienza, ad un impegno costante e preciso verso la pace, sembrano essere un bersaglio facile di atti di crudeltà e di vera cattiveria, tanto da essere iscritti come vere e proprie persecuzioni contro la libertà di parola, di espressione e di culto. Purtroppo, davanti a noi tutto ciò e questo lo dobbiamo sottolineare con particolare attenzione rispetto alle giovani generazioni - appare nell'opinione pubblica occidentale un aspetto quasi marginale. C'è una sorta di disattenzione. Sembra quasi che l'opinione pubblica non sia interessata a tutto ciò.

Anche in Europa la cultura dominante preferisce muoversi con estrema cautela, ma questo rischia di far smarrire quel senso di appartenenza alla nostra storicità cristiana, viva e forte in Europa È come se ci si vergognasse di noi stessi, delle nostre tradizioni di civiltà ed uguaglianza, delle conquiste umane e sociali, e quindi ricacciamo la conoscenza di questi soprusi in fondo alla nostra coscienza, e comunque sempre nelle ultime pagine dei nostri quotidiani. Eppure, la libertà di parola, di espressione e di culto, sono diritti che continuano ad essere ampiamente violati. Sono e continuano ad essere la base giuridica della nostra Costituzione e delle nostre moderne costituzioni.

con gli altri Stati, ha sempre posto nell'agenda degli incontri politici il tema dell'uccisione dei cristiani nel mondo. Anche le Nazioni Unite, attraverso l'Alto commissariato per i rifugiati,

cerchi di combattere ogni forma di incitamento all'odio contro tutte le comunità religiose e non abbassi assolutamente la guardia rispetto alla persecuzione dei cristiani nel mondo. Infine, proprio perché la preoccupazione è quella della conoscenza per non dimenticare, chiediamo al Governo che nelle Commissioni parlamentari competenti annualmente un rapporto sullo stato delle persecuzioni avvenute nel mondo per tutti i motivi religiosi. *(Applausi

alle persecuzioni per motivi religiosi, pensando che il tema fosse più ampio di quello incentrato solo sulle persecuzioni anticristiane.

è ancora oggi in preda a sommovimenti di straordinaria profondità ed estensione, per cui riesce un po' difficile parlare soltanto delle persecuzioni anticristiane. Ci convince di più riferirci ad un contesto più vasto. Vorrei provare a a sottolineare la natura complessa e dialettica di tale argomento, perché non è facilissimo tracciare un confine di identità preciso sulla persecuzione religiosa. Nella storia dell'uomo le persecuzioni religiose sono intrecciate in modo inestricabile con una logica di appropriazione, di stravolgimento, di dominazione

qualche volta ha avuto una funzione ancillare, altre volte è stata utilizzata come mero strumento dalla politica. davvero difficile stabilire un confine preciso. Quando ci interroghiamo sugli scontri tra identità sociali, etniche, nazionali, nazionalistiche e religiose, è assai difficile riuscire a stabilire una distinzione tra quale sia l'elemento decisivo, quello trainante e quello trainato. Non ho il tempo di trattare gli infiniti esempi che la memoria storica ci riserva, ma fin dalla

cristiani possedessero una straordinaria capacità nella sottomissione e nel massacro degli indios, tanto che questi furono ridotti in poco più di mezzo secolo da circa

così ci racconta la storiografia - ad immaginare una variazione profonda della legislazione nei confronti della condizione degli indios.

che qualche decennio dopo, alla fine del '500, rifletteva sulle tragedie della sua società, va continuamente con la memoria - che è poi quella dell'attuale, del recente - alla straordinaria disgrazia delle guerre di religione,

scontri, incontri e separazioni. Si potrebbe essere sedotti da un'idea, quella cioè che gli Stati nazionali abbiano favorito una sorta di istituzionalizzazione della religione, per cui su quella base, o anche su quella base, sono state esercitate delle separazioni. Se si fa un'analisi delle società mediterranee

interetnici, interculturali, interreligiosi siano a poco a poco stati ridotti a unità dalla prevalenza di un soggetto sull'altro. A Cipro, turchi e greci convivevano, forse non in modo idillico, ma, per impulso dei colonnelli greci, negli anni '50 del Novecento si è determinata una separazione netta: la capitale fu spaccata, turchi e greci stavano in parti diverse e così via. Non è il caso di eccedere in pedanterie narrative, ma la storiografia che ha riflettuto su questi argomenti è abbastanza concorde nell'ammettere che un uso politico della religione o una volontà politica di utilizzare la religione come strumento ha facilitato più la separazione che il dialogo, più la fissazione di limiti tra gruppi umani che la loro interrelazione. È il costituzionalismo recente, recentissimo, che sa immaginare un altro destino. Ma noi in realtà da questo punto di vista siamo abbastanza all'alba di una nuova condizione: lottiamo contro determinismi molto radicati, affondati nella tradizione, e incontriamo anche molte difficoltà a fronteggiarli. Il nostro mondo mediterraneo circostante è stato fino a poco tempo fa dilaniato da fenomeni di questo tipo. I bosniaci sono tornati ad essere islamici, mentre lo erano molto meno prima, perché hanno lottato contro i serbi ortodossi. C'è una complicazione immanente di fronte a noi e, di fronte a questa complicazione, la parola del costituzionalismo moderno è che invece bisogna perseguire le ragioni del dialogo, dell'interrelazione e della tolleranza. Tutte le parole sono ambigue. Gli illuministi che avevano inventato la tolleranza hanno anche loro praticato lo schiavismo. In effetti, la materia è molto sfuggente. Pur con la consapevolezza che la materia è effettivamente

costituzionalismo - davvero recentissimo - rappresenta una via maestra per affrontare problemi che nessuno potrà cancellare e che continueranno ad essere di fronte a noi. Per questo motivo, la nostra nostra mozione tende a impegnare il Governo a mettere in atto ogni utile iniziativa diplomatica al fine di contrastare con efficacia i soprusi perpetrati, in ogni angolo del mondo, a danno di uomini e donne di ogni razza o etnia, a causa della professione del loro credo religioso.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, più che mozioni noi avremmo dovuto proporre oggi in Aula interrogazioni, poiché, non più tardi di un anno fa, noi abbiamo qui discusso della situazione dei cristiani perseguitati in diverse parti del mondo, fino a giungere a un ordine del giorno condiviso che impegnava il Governo ad assumere iniziative sul piano internazionale. Se la voce del Senato della Repubblica e la sua volontà non sono vane, dovremmo oggi ricevere dal Governo risposte puntuali sull'atto approvato il 30 ottobre 2008. Voglio dire che la realtà di cui stiamo parlando è troppo seria perché essa possa essere periodicamente evocata nello spazio libero e un po' vuoto dell'Aula. Torniamo dunque oggi sui fatti che sono noti, registrando purtroppo altri episodi di violenza e intolleranza etnica e religiosa. Per tutti, cito due fatti recenti: quello avvenuto a Gojra, nel Punjab orientale, in Pakistan, quando, nei primi giorni dell'agosto scorso, centinaia di estremisti musulmani hanno aggredito e arso vivi alcuni cristiani, tra i quali quattro donne e un bambino, accusati di aver profanato il Corano in occasione di una festa nuziale.

del *Lord's Resistance Army*, gruppo armato nato nell'Uganda del Nord e responsabile di attacchi contro civili nell'area tra Sudan, Repubblica democratica del Congo e Uganda, hanno fatto irruzione nella chiesa di Nostra Signora della Pace nella città di Ezo, hanno rapito alcuni ragazzi tra i 15 e i 20 anni e ne hanno uccisi sette, crocifiggendoli. Questo è il nostro mondo, il mondo di oggi. Guardiamo all'Africa, soprattutto, dove forse più acuto è il dramma delle guerre, delle violenze tra etnie e delle persecuzioni nei confronti di comunità cattoliche, e dove la gente dei villaggi è costretta alla fuga e in balia ai ribelli armati. L'Africa di oggi, che si affaccia al mondo con le sue grande potenzialità, ma anche con le sue ferite profonde, chiama in causa noi e il mondo intero, chiama in causa l'Unione europea alcuni decenni dopo il colonialismo, mentre interessi economici e politici dall'Europa e dal resto del mondo tuttora tentano di condizionarne lo sviluppo economico e politico. L'Africa chiama in causa l'ONU, presente ma impotente nei luoghi dei conflitti africani. Se la politica internazionale non agisce con determinazione e lungimiranza, avendo come interesse prioritario la giustizia e la pace, continueremo a registrare, soprattutto in Africa, il perdurare dei conflitti tra etnie e religioni, spesso paravento di interessi economici e di potere. Continuerà a pagare la società civile, pagheranno le donne e i bambini, vittime della violenza e delle sopraffazioni che la politica non sa fermare. Non basta denunciare: occorre che la politica si impegni. È per questo che, ancora una volta, chiediamo al Governo di agire nel contesto internazionale affinché sia posta fine ai conflitti e ai focolai di violenza. che l'Unione europea, insieme all'ONU, non possa intervenire sul piano politico e diplomatico perché siano portati a soluzione i conflitti nel Nord Kivu e nel Sud Kivu? Come non comprendere che per fermare le persecuzioni dei cristiani non basteranno gli appelli ma sarà necessaria una credibile azione politica dell'Unione europea, degli altri grandi Paesi del mondo, della Cina e dell'ONU? Quest'azione, finora, è stata sin L'azione che, su questo terreno, ha di recente iniziato a svolgere in Africa Romano Prodi per incarico del Segretario generale delle Nazioni Unite è il segno di uno sguardo di più lungo orizzonte, per un'assunzione di responsabilità più profonda, sia dell'ONU, che dei Paesi africani e della stessa Unione africana. La voce di quest'Africa si è levata con forza nella seconda Assemblea del Sinodo per l'Africa, svoltosi a Roma l'ottobre scorso. In quell'occasione il cardinale di Khartoum, Zubeir Wako, ha detto: «L'Africa ha bisogno di pieno rispetto e l'Africa deve darlo a se stessa». Nell'Assemblea del Sinodo africano, non è solo la Chiesa africana che ha parlato a Roma, ma è la Chiesa universale che si è riunita a Roma per riflettere sulla situazione del continente africano. La storia ha posto l'Italia e la sua capitale nella condizione privilegiata di sentire in modo molto ravvicinato il grido di dolore e di speranza che viene da quel Continente. È una responsabilità in più per noi, abbiamo sentito da vicino la Chiesa africana denunciare il disprezzo per i diritti umani, la mancanza di libertà, la politicizzazione della religione come male diffuso, anche se in misura differenziata, nelle 53 Nazioni africane, mentre la stessa Chiesa ha riconosciuto il bisogno di diventare una Chiesa riconciliata, dopo aver attraversato anch'essa i massacri del Continente. Non dobbiamo soltanto registrare i fatti, ma dobbiamo capire ed interpretare i processi. La politica è interpellata in modo radicalmente nuovo nel mondo globale, e la comunità internazionale non può affrontare in modo frammentato i problemi del mondo: se vogliamo agire efficacemente per fermare le violenze e le persecuzioni a causa della religione, dobbiamo cercare modelli più avanzati di integrazione e di dialogo interculturale ed interreligioso, e più estesi strumenti di solidarietà e di cooperazione tra i popoli. Significa lottare contro la discriminazione, il razzismo, la xenobia, il fondamentalismo religioso che considera l'altro di diversa religione un nemico; significa imparare che la civiltà - come sempre è accaduto nella storia, a tutte le latitudini - è mescolanza di diversità e che le religioni possono e debbono convivere e dialogare nel rispetto reciproco, promuovendo umanità, solidarietà, sviluppo potremmo aggiungere, democrazia e pluralismo. Abbiamo imparato nei secoli anche noi in Europa che l'uso strumentale e politico della religione genera guerre; abbiamo imparato che la ragione e la laicità sono un presidio per il rispetto della vita e della dignità dell'uomo. Questo è il patrimonio che oggi dobbiamo consegnare e seminare nel mondo. Proprio sul dialogo interreligioso, la proposizione n. 11 del Sinodo della Chiesa africana è esplicita: «Il dialogo con le altre religioni, specialmente l'Islam e la religione tradizionale africana, è parte integrante della predicazione del Vangelo». Colleghi, tutto ciò riguarda anche noi oggi in Italia. Il riconoscimento e il rispetto della libertà religiosa, del dialogo interreligioso ed interculturale - anche in Italia - non è mai una conquista per sempre, mentre resta parte dell'orizzonte universale del mondo nuovo che stiamo costruendo. Non si è spenta l'eco - e credo che durerà a lungo - dell'attacco rivolto nei giorni scorsi all'Arcivescovo di Milano da parte di un Ministro del Governo italiano e del giornale del suo partito. Una miscela di ignoranza, arroganza del potere, calcolo strumentale di convenienza politica, ha colpito il Cristianesimo nella sua essenza, l'annuncio del Vangelo, sotto il cielo di Milano, ma sotto tutti i cieli, poiché le parole dei vescovi africani e del cardinal Tettamanzi sono esattamente le stesse. Il Presidente della Repubblica ha dato voce al nostro popolo, dicendo che il ruolo della Chiesa, dei suoi valori spirituali e culturali è essenziale per la società italiana». Il patto costituzionale della Nazione e la stessa dignità della politica si fondano sul rispetto reciproco. Con questa consapevolezza, chiediamo oggi al Governo di farsi interprete nel mondo della vocazione dell'Italia per la pace, per il dialogo e per la libertà religiosa, sapendo che saremo credibili solo se per primi realizzeremo questi valori nel Il rispetto che chiediamo oggi per i cristiani in Africa e nel mondo è lo stesso che invochiamo per ogni persona, qualunque sia la sua religione. Abbiamo davanti agli occhi il numero sterminato delle vittime di ogni violenza a causa della libertà, compresa quella di religione; abbiamo davanti agli occhi le popolazioni sterminate che girano per il mondo e arrivano anche in Italia con i loro diritti universali, che una società moderna e costituzionalmente democratica deve saper rispettare ed interpretare. Questo ci dice oggi l'universalità del Cristianesimo. Questo ci dice la dignità della politica: sentiamone la responsabilità. La nostra Costituzione, pagata a così caro prezzo,

una nuova finestra"). Sono presenti in tribuna gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «Giacinto Dell'Olio» di Bisceglie, in provincia di Bari. A loro rivolgiamo il nostro saluto e gli auguri per la loro attività di studio.

dei cristiani nel mondo. Un anno fa si parlò dell'India, oggi si è parlato - ma fortunatamente si è avuto anche modo di ampliare la questione nell'illustrazione dei documenti - del contesto africano.

sul suolo patrio, non del tutto estranee al dibattito che stiamo svolgendo oggi. Infatti, se è vero - come è vero - che i cristiani sono il gruppo religioso maggiormente perseguitato nel mondo, è altrettanto vero che sono l'unica organizzazione religiosa nel mondo che siede in quanto tale all'Assemblea generale

delle loro manifestazioni) e sono stati malmenati dalla polizia e dall'esercito. Spero che si possa tenere in considerazione anche questo contesto drammatico che non è in Africa.

La senatrice Soliani si è più volte appellata alla necessità di essere attivi nel contesto internazionale. Rielaborando tutto il suo intervento, credo che la parola chiave sia stata «responsabilità». L'Italia da sempre è capofila capofila per quanto riguarda le mobilitazioni e il rispetto dei diritti umani: forse più all'estero che a casa propria (mi riferisco in particolare alla campagna mondiale per l'applicazione di una moratoria universale sulla pena di morte),

cittadini di Paesi africani verso cui l'Italia può effettivamente prendere in considerazione richieste di *status* di rifugiato, vi sono nigeriani, eritrei, sudanesi che, proprio da luoghi dove il Cristianesimo non può essere praticato, fuggono da soli o con le proprie famiglie. L'ultimo impegno che la mozione del PD che ho sottoscritto

che ancora oggi, malgrado la legge imponga che sia fornita loro una risposta entro 35 giorni, si trovano nel più totale limbo. Ebbene, il limbo è stato abolito dalla Chiesa cattolica. Noi crediamo debba essere abolito anche dal Governo italiano per quanto riguarda il rispetto dei trattati internazionali. Concedere una protezione di qualsiasi tipo a chi fugge da una persecuzione religiosa deve essere uno degli impegni con cui il Governo oggi esce da questo dibattito d'Aula, che abbiamo voluto si svolgesse non per occupare del tempo, ma per discutere di un problema gravissimo nel mondo.

avviene la maggior parte delle persecuzioni, come una sorta di colonialismo culturale. Tuttavia, questa visione forse ancora diffusa, magari anche nelle nostre scuole, è completamente

effettivamente essere ripreso e portato all'attenzione dell'opinione pubblica.

delle stesse. Certo, non si parla di problemi di persecuzione ma credo che questa occasione sia opportuna per ricordare che, anche al nostro interno, dobbiamo cercare di dare il buon esempio e farci promotori, proprio perché sappiamo quel che è successo in Europa per tanti secoli e quindi abbiamo l'esperienza e la credibilità necessarie per rivolgere un appello davvero forte e per essere incisivi e chiari, mostrando di non essere disposti a passi indietro, a chiudere un occhio o tutti e due, in particolare con i Governi di Paesi in cui questi episodi di persecuzione gravissima avvengono.

quello che colpisce secondo una ricostruzione credo attendibile è che nell'arco di 2.000 anni sarebbero stati

quindi conosciuto negli ultimi tempi della nostra storia universale un'accelerazione gravissima. Sono oggi 60 i Paesi che manifestano una condizione per la quale si può parlare di una vera e propria persecuzione. Nel corso del tempo, soprattutto soprattutto del Novecento, ideologie contrapposte ma unificate attorno ad una visione atea del mondo hanno avuto una comune

qualcosa che annuncerà la fine del mondo, vi sarà una persecuzione che riguarderà i cristiani. «Prima di tutto questo» - avverte il Signore - «metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno». I cristiani sono dunque pronti e sanno che la persecuzione è nell'orizzonte della loro testimonianza di fede. Ma il martirio - questo è interessante da un punto di vista laico, laico, e lo ha precisato bene l'allora cardinale Ratzinger in un suo intervento - è la «capacità di verità dell'uomo quale limite di ogni potere e garanzia della sua somiglianza divina». Noi dobbiamo attenerci a questo. Il martirio è una risposta nei confronti di un potere che presume di poter disporre dell'uomo. Oggi la reazione del Cristianesimo e dei cristiani, fortunatamente e giustamente, non è una reazione armata. Non siamo ai tempi delle crociate. Quindi, possiamo individuare come questa evoluzione consenta di inquadrare la risposta nei termini più corretti e giusti, cioè come una capacità di accogliere le diversità, anche le difficoltà estreme, in un contesto fatto di dialogo, soprattutto difficile, ma importante, come quello religioso. Oggi le violenze, colleghi, sono prevalentemente nascoste dietro il manto della religione, ma spesso portano qua e là alla luce problemi di fondo, problemi che attengono all'organizzazione del potere. Basti citare il caso dall'India dove la testimonianza cristiana, in realtà, mette in crisi l'assetto per casta della società indiana

in quanto tale; se non c'è libertà, non c'è neanche la condizione per la giustizia, sia all'interno di un contesto nazionale sia a livello internazionale; e se non c'è giustizia, non c'è neppure pace. Non a caso, poco più di un mese fa, il Dipartimento di Stato di Washington, nel presentare il rapporto annuale sulla libertà religiosa nel mondo, ha rilevato come sia necessario evitare che si radicalizzino gli scontri religiosi, che hanno per conseguenza, appunto, un'oppressione nei confronti di alcuni particolari gruppi religiosi, in modo particolare quelli legati alla fede cristiana. «D'altra parte», si legge nelle ultime righe dell'introduzione a questo rapporto, «un ambiente di salda libertà religiosa promuove l'armonia nella comunità e rafforza le voci moderate apertamente si oppongono agli estremisti attraverso motivazioni religiose»; quindi, combattere contro le persecuzioni significa combattere contro tensioni nascoste o palesi che possono mettere in discussione la condizione di equilibrio e di sicurezza internazionale. Vorrei aggiungere, colleghi, che lottare contro l'intolleranza e le persecuzioni vuol dire compiere ulteriori passi avanti verso la civilizzazione mondiale. L'Europa ha imparato, negli ultimi due secoli, ad aprirsi alle altre culture e alle altre religioni. Il grande storico Toynbee sosteneva che l'incontro dell'Occidente con il buddismo avrebbe costituito «l'evento

di aprire noi stessi, nel momento in cui chiediamo agli altri di aprirsi e di rispettare i diritti fondamentali dell'uomo, innanzi tutto il diritto a professare la libertà di culto. Ecco perché, come ha ricordato la collega Soliani, è sbagliato chiudere in un involucro di protesta e di accidia la questione dell'integrazione tra comunità diverse all'interno della nostra Nazione; è sbagliato l'attacco al cardinal Tettamanzi; è sbagliato chiedere a noi stessi una cosa diversa rispetto a quanto chiediamo alle altre Nazioni. In questo spirito, noi impegniamo il Governo non solo affinché riferisca stabilmente, cosa che non ha fatto nel corso dell'ultimo anno nonostante la mozione dell'ottobre scorso, ma soprattutto perché sviluppi un'iniziativa diplomatica, in sede di grandi organizzazioni internazionali - all'interno dell'ONU e della Comunità europea - perché questi principi costituiscano l'intelaiatura non di affermazioni sporadiche ma di una politica stabile che valorizzi fino in fondo il genio, la caratteristica, la sensibilità,

splendida trattazione la collega Laura Bianconi e al quadro che si è formato durante questo dibattito per proporre un approfondimento, come cofirmatario della mozione n. 194, nella direzione ancora una volta delle responsabilità. Lo faccio come vice presidente della Commissione che in Senato si occupa di politiche dell'Unione europea, perché da adesso in poi l'Europa non può più nascondersi. L'assordante silenzio - per usare una metafora abusata - dell'Europa finora su questo scenario mondiale, dove si sono perpetrati questi orrendi delitti, non ha più un alibi. Da otto giorni è entrato in vigore il Trattato di Lisbona, che attribuisce all'Unione europea reali poteri di politica estera ha creato per questo un vero e proprio Ministro degli esteri, pomposamente reclamizzato. Mi rivolgo al sottosegretario Mantica affinché sia latore del seguente messaggio: ci attendiamo che questa grande innovazione portata dal Trattato di Lisbona si traduca in iniziative concrete, ora possibili, non tanto e non solo nei confronti dei gruppi di ribelli che sono autori di questi efferati delitti ma dei Governi, che forse in maniera troppo rassegnata non si attivano per combatterli e contrastarli. Vorrei ricordare che l'Unione europea, finora, non è stata totalmente assente da questi scenari, ma era presente con le politiche per la cooperazione e lo sviluppo con gli aiuti umanitari elargiti in maniera davvero davvero consistente in tutti i 60 Paesi qui indicati come teatro di questi efferati delitti. Quindi, l'Europa poteva intervenire; è stata presente, ma con le mani legate: non avendo poteri di politica estera certamente non avrebbe potuto, e non lo ha fatto, interloquire con i Governi responsabili di troppa rassegnazione. Ora lo può fare, e lo può fare anche concretamente, sottosegretario Mantica, magari utilizzando quei 15 gruppi tattici che l'Unione europea ha costituito molti anni fa, forti da 1.500 a 3.000 uomini, che non sono stati quasi mai impiegati, laddove invece avrebbero dovuto essere inviati in focolai di crisi regionali e soprattutto di disordini, come quelli di cui si parla in queste mozioni. Non è più il tempo degli alibi per l'Europa. Anche i vescovi, in due riprese molto ravvicinate, come è stato ricordato dai colleghi, hanno ora il coraggio di puntare il dito contro contro l'Europa. Lo hanno fatto in maniera esplicita anche a Roma nel mese di ottobre, e prima ancora in Africa; chiedono, come dice anche la nostra mozione, all'Europa ed a tutta la comunità internazionale di guardare con più attenzione e di intervenire in maniera più concreta. Si può fare: oggi dobbiamo farlo. Diceva la collega Soliani che l'ONU è stata presente ma impotente; direi che l'Europa è stata impotente perché assente.

scambio, di affari e di cooperazione, a vari livelli; ebbene, signor Sottosegretario, incominciamo a condizionare tale presenza e la stesura e la firma di tali rapporti al rispetto di queste libertà. Nella nostra si dice che il diritto alla libertà religiosa è un elemento che bisogna garantire ad ogni persona, così come la libertà di parola e di espressione. Quindi, la prego di aggiungere alle molte proposte che oggi che oggi ha raccolto e raccoglierà anche quella di dare una scossa elettrica all'Europa; ora non ha più le mani legate, deve solo imparare ad usarle, affinché quell'assordante silenzio non divenga una clamorosa colpa di tutti noi.

Presidente, il compito del Governo non è facilissimo, perché apparentemente le tre mozioni trattano lo stesso argomento; in realtà, come si evince dalla discussione generale e da quanto

apparentemente molto semplice, ma che in realtà è estremamente complesso proprio per le molte chiavi di lettura che ruotano attorno a questo principio.

Al riguardo bisognerebbe fare un approfondimento perché i casi citati corrispondono anche a situazioni in cui la religione è strumento di lotta politica. Quando parliamo di India, affermiamo che la religione cristiana elimina le caste e ciò provoca le reazioni degli indù e dei musulmani nella misura in cui il Cristianesimo, nella sua concezione legata alla persona, supera il concetto di casta, che a a noi non piace, ma che è ancora una delle strutture portanti dell'organizzazione sociale indiana e, quindi, è un attacco alla libertà religiosa collegato strettamente ad una realtà sociale di quel Paese.

abbiamo posto all'ordine del giorno il problema degli atti di violenza contro le persone appartenenti a minoranze religiose, indicando nella difesa della libertà di religione non tanto una difesa del Cristianesimo quanto la difesa di un principio che è fondante dell'Unione europea. europea. Pertanto, se l'Unione europea non si fa garante e non si pone in prima fila nella lotta contro le discriminazioni delle minoranze religiose tradisce uno dei suoi elementi fondanti. Nella riunione del 16 novembre scorso è stata approvata una risoluzione da parte dell'Unione europea sotto la Presidenza svedese, in cui sono state ribadite la centralità del tema della difesa delle delle minoranze religiose nella politica estera dell'Unione europea e l'intenzione di considerare ulteriori iniziative per promuovere l'azione a favore della libertà È importante sottolineare i due aspetti alla base di questa presa di posizione: da un lato, la volontà di riaffermare all'esterno questo principio, che delinea e definisce una delle caratteristiche dell'Unione europea;

incluse quelle cristiane, e richiama gli Stati nazionali ad un maggiore impegno per arginare questi fenomeni. Il testo è stato approvato per consenso dalla Terza Commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dovrà essere successivamente ratificato dall'Assemblea plenaria. avviso, si tratta di un primo, piccolo ma significativo risultato: infatti, dobbiamo dire apertamente che non è stato facile coagulare il consenso di tutti gli Stati su un tema come questo, sul quale esistono sensibilità differenti,

È intenzione del Governo continuare a mantenere in tutte le sedi il tema al centro dell'azione nel campo dei diritti umani, lavorando all'interno dell'Unione europea affinché questa sappia assumere una posizione responsabile, ma soprattutto trovare i mezzi per essere in grado di reagire prontamente

Governo a proseguire nelle iniziative diplomatiche, chiarendo quindi che non si comincia da oggi questo tipo di attività: questa mozione serve anzi a rafforzare le iniziative finora assunte, così

motivo per non essere d'accordo con lei, ma vuole solo ricordare che l'Unione europea ogni anno pubblica un Rapporto annuale sui diritti umani, all'interno del quale è presente un capitolo che illustra quanto questo organismo fa per

vorrei ricordare che quest'ultimo si presenta come il portavoce di Dio, *medium* dello Spirito Santo e figlio della Madonna. Il problema non è evidentemente che lo si accusa di essere un estremista cristiano o di essere un estremista religioso.

Vorrei ricordare che l'LRA e i suoi dirigenti sono stati incriminati dalla Corte penale internazionale per avere attuato violazioni dei diritti umani compresi omicidio, rapimento, mutilazione dei genitali, riduzione in schiavitù sessuale di donne e bambini, costringendo tra l'altro i bambini stessi a partecipare alle ostilità come bambini soldato. l'altro, che l'LRA nei suoi metodi di arruolamento dei bambini prevede l'uccisione dei genitori da parte dei bambini arruolati proprio per creare la frattura con la realtà del villaggio e con il mondo tribale.

modo, in Etiopia non risultano particolari movimenti di violenza incentrati sulla libertà religiosa che la Costituzione etiopica è una delle poche Costituzioni africane a prevedere la libertà di religione - siamo a livello di scontri tra musulmani e cristiani ortodossi. Vorrei rispondere al senatore Malan, che ha parlato di un aumento dei cristiani in Africa,

se per Cristianesimo si intende la religione cattolica o quella protestante, francamente mi sentirei di discutere su questo incremento. Parlo di sette perché naturalmente procedono

anche perché l'Eritrea purtroppo per noi è diventata recentemente un terminale dell'Iran per la distribuzione delle armi in tutte le zone di contestazione e di guerriglia all'interno delle realtà africane.

A legislazione vigente possiamo assumerci l'impegno di continuare a dar seguito alle procedure di riconoscimento e al diritto all'asilo.

Ritengo di aver espresso un parere sostanzialmente positivo con queste piccole correzioni, che sono peraltro integrative di un'azione che il Governo continua a svolgere da tempo. Ribadisco che il Governo ritiene che, nel campo dei diritti umani, un'azione prioritaria da svolgere, come ha già fatto in sede di Assemblea generale dell'ONU e in sede di Conferenza generale dei Ministri degli esteri il 16 novembre a Bruxelles. Il Governo ringrazia pertanto tutti gli intervenuti e continuerà a mantenere i propri impegni.

Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, nei classici di storia delle dottrine,

Non è un caso, a mio avviso, che questo processo si sia compiuto negli stessi anni in cui si sviluppava un'idea sbagliata della libertà religiosa, intesa più come tolleranza reciproca che come rispetto; più come ricerca di soluzioni sincretiche che non come esaltazione delle differenze. Tutto ciò ha portato a un progressivo smarrimento che le religioni non coincidono con le culture: le culture si contaminano, cambiano, si modificano con il tempo;

E solo il rispetto della propria fede suscita nelle altre religioni un atteggiamento di rispetto nei confronti della fede degli altri. Come ha detto bene Benedetto XVI, in questa dinamica le religioni si rafforzano a vicenda.

né una richiesta di carattere sindacale o di tipo corporativo. Dal dibattito di stasera abbiamo appreso che la reciprocità è, innanzitutto, un'azione contro la violenza. Nutrire e pretendere rispetto per la propria fede, per la fede dei propri padri, indipendentemente dal fatto che si creda o meno,

quindi che vada salutato con grande soddisfazione questo dibattito, che è un altro piccolo ma concreto segno di un'inversione di tendenza.

ci si è resi conto nuovamente dell'importanza di questo fattore nel dibattito pubblico. Oggi constatiamo che abbiamo meno complessi nel denunciare le persecuzioni religiose e la violazione del principio della libertà religiosa. non dobbiamo avere remore nel parlarne e nel farne oggetto di comunicazione e di sensibilizzazione. In caso contrario, colleghi senatori, oscurando le persecuzioni ai danni dei cristiani nel mondo rispetto ad analoghi episodi perpetrati nei confronti di appartenenti ad altre confessioni religiose, si rischia solo di alimentare il sentimento di rifiuto e di rivalsa rispetto alle altre religioni. Ed è quello che non vogliamo che avvenga. Affrontare questi drammi, maturare piena consapevolezza e intraprendere tutte le azioni politiche possibili affinché non si ripetano più, è il modo migliore per affermare che la libertà religiosa è un principio inviolabile per tutti e nei confronti di tutti.

Queste mozioni non sono ovviamente, nemmeno lontanamente, di censura. Vogliono piuttosto essere mozioni di stimolo, tese a creare quella unità necessaria tra Governo e maggioranza, perché su temi di questo tipo essi non devono trovarsi in una condizione di dialettica, ma piuttosto descrivere un *continuum*. Perché, signor Presidente, se si è timidi nel denunciare ciò che accade nei confronti della religione che ha scritto pagine importanti della propria civiltà, poi non ci si può stracciare le vesti di fronte ad episodi come il *referendum* svizzero, che tradiscono non il rifiuto dell'altro, quanto un bisogno di rispetto che non sempre le classi politiche riescono ad interpretare. Io credo che, anche in questo caso, dei segni importanti siano venuti persino dalla comunità musulmana. Ho letto con interesse le dichiarazioni del portavoce della moschea di Brescia che, riferendosi a quel risultato, ha affermato

interpretato naturalmente in modi e con sensibilità diverse. In fondo, però, c'è un richiamo comune che è un segno positivo che vogliamo sottolineare. È per questo motivo che il Gruppo del PdL voterà favorevolmente a tutte e tre le mozioni.

firmata in maniera trasversale da tutti i Gruppi politici, il problema nei confronti di comunità cristiane nel mondo è universalmente sentito. Noi dell'Italia dei Valori siamo i primi a condannare le efferate torture che i cristiani subiscono nei vari angoli del pianeta. Pensare che nel terzo millennio seguire le proprie convinzioni religiose possa significare la morte non è accettabile. Come ben saprete, cari colleghi, alcuni Stati portano avanti una politica di repressione nei confronti dei movimenti religiosi o spirituali non autorizzati. Siano i fedeli cristiani, musulmani, ebrei o buddisti, la persecuzione in alcuni Paesi minaccia la loro fede e mette a repentaglio la loro vita. io sono convinto che nessuno Stato abbia il diritto di mettersi in una posizione tale da dettare legge su questioni attinenti alle coscienze individuali. La libertà di culto dovrebbe essere garantita in ogni Stato del nostro pianeta. Finché questo non avviene, noi abbiamo il dovere proteggere tutte quelle persone che desiderano professare liberamente il proprio credo, sempre nel rispetto del prossimo. Il 14 settembre di quest'anno si è aperta a Ginevra la XII sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Nel suo discorso di apertura, l'Alto Commissario ONU per i diritti umani ha delineato i settori critici sui quali le Nazioni Unite dovrebbero intervenire. Noi siamo perfettamente d'accordo nel tutelare le vittime civili di guerre e nel cercare di ridurre le eccessive differenze economiche che dividono le persone e le aree del nostro pianeta, ma ci sarebbe piaciuto vedere contemplato, nell'agenda del Consiglio, il problema dello stillicidio quotidiano di vittime perseguitate, torturate e uccise per motivi religiosi. Concentrando la nostra attenzione sui fedeli cristiani, il problema della persecuzione non è inesistente, anzi, viste le cifre, dovrebbe essere affrontato anche con maggiore specificità. vorrei farvi fare un piccolo, e ovviamente virtuale, giro del mondo per farvi capire l'entità del problema. Partirei proprio dalla Cina. In questo Paese tutte le religioni sono illegali. Come forma di culto è ammessa solo l'adorazione verso il partito comunista. Cristiani, islamici, buddisti non hanno il diritto di professare liberamente il loro credo. La politica di repressione nei confronti delle comunità cattoliche nella Repubblica popolare cinese ha avuto inizio durante la guerra civile del 1947. Le guardie di Mao, all'epoca, assalirono numerosi monasteri, picchiando e torturando monaci trappisti e suore. Mao considerava i cattolici "i nemici senza fucile" e ordinò l'arresto di migliaia di credenti. Tornando al 2009, possiamo dire che la politica di ieri è ancora la stessa del Governo di oggi. Il culto dello Stato viene imposto attraverso la sistematica lotta contro le altre fedi. I cristiani, cattolici e protestanti, vengono ancora considerati agenti delle potenze straniere e per questo motivo esponenti religiosi, ma anche fedeli, sono vittime di incarceramenti, pestaggi e torture. Per contrastare la Chiesa cattolica, il Partito comunista, nel 1957, ha creato la Chiesa patriottica cinese, l'unica ufficialmente accettata. L'autorità della Santa Sede non viene accettata e vescovi e sacerdoti vengono scelti tra i nominativi graditi al Partito. La vera Chiesa è clandestina ed è continuamente oggetto di attacchi. I «Regolamenti per le religioni», introdotti nel 1994, impongono a tutte le comunità religiose di registrarsi presso l'Ufficio affari religiosi, che controlla e sostanzialmente impedisce il lavoro dei missionari e la pratica religiosa dei fedeli. Vengono infatti imposti i ritmi con i quali professare i riti e viene stabilito a tavolino, dai funzionari del partito, il programma da insegnare nel catechismo. Vescovi e sacerdoti sono continuamente indagati e controllati dalla polizia ed alcuni di loro sono recentemente spariti. Oggi si assiste poi ad un nuovo fenomeno. Le autorità cinesi, infatti, guardano con preoccupazione il riavvicinamento che ha interessato alcune frange della Chiesa patriottica alla Chiesa cristiana. Nonostante tutte le vittime che la repressione cattolica cinese ha provocato, il numero dei cristiani è aumentato e, di conseguenza, è incrementato anche il numero di individui potenzialmente soggetti a persecuzioni e che, dunque, andrebbero tutelati. Ma i cattolici rappresentano solo una delle comunità religiose minacciate. Nel 2007 il Governo cinese ha avviato una campagna contro le comunità protestanti e il 13 settembre di quest'anno a Linfeng, nello Shanxi, 400 poliziotti hanno compiuto, proprio in nome di questa campagna, un raid notturno contro una cappella protestante situata all'interno di una fabbrica di scarpe. L'edificio è stato abbattuto, la chiesa è stata ridotta in macerie, i mobili e i soldi contenuti nella struttura sono stati rubati, ma ancora più gravi sono state le violenze fisiche che hanno dovuto subire i fedeli accorsi e l'ordine di non soccorrere i feriti imposto ai medici dell'ospedale della cittadina. Numerosissimi esempi di altrettanto gravi episodi possono purtroppo essere fatti anche riguardo la persecuzione dei buddisti. Al di là dei danni strutturali che vengono inferti ai monasteri tibetani, trovo sconvolgente una cifra: da 100.000 monaci buddisti inizialmente operanti nel Paese, ne rimangono oggi solo 6.000. Monaci e suore tibetani vengono continuamente picchiati, incarcerati e rapiti. La stessa efferatezza colpisce inoltre i musulmani cinesi. La popolazione, in seguito al tristemente famoso massacro del 1997 e a numerosi e continuativi attacchi mortali, è ridotta oggi quasi alla metà di quel che era un paio di decenni fa. Sono dati sconvolgenti, ma l'opinione pubblica è già al corrente in parte della repressione portata avanti dal Governo cinese nei confronti delle comunità religiose. Meno note sono invece quelle situazioni di rischio che interessano le comunità cattoliche residenti in altri Paesi. In Arabia Saudita il 3,7 per cento della popolazione è di fede cristiana e costituisce il gruppo non musulmano più numeroso e più organizzato: si stima siano intorno ai 900.000. Nel Regno saudita, dove la libertà religiosa non è contemplata, i gruppi di preghiera cristiani divengono, quindi, il bersaglio preferito dalle autorità del Regno. Negli ultimi anni episodi di efferatezze, torture e arresti sono stati all'ordine del giorno e dal 1985, anno di espulsione dell'ultimo sacerdote cristiano, nel Paese non risiedono più né sacerdoti, né religiosi. Il problema principale è che la politica e la religione sono un tutt'uno, e spesso l'accusa di professare il credo cristiano viene usata per annientare i dissidenti politici del regime. In Arabia Saudita, come del resto avviene in quasi tutti i Paesi musulmani dove vige la *Sharia*, non è contemplata la possibilità di conversione, e chiunque desideri incontrare una fede religiosa diversa da quella musulmana rischia, per legge, di essere condannato a morte e giustiziato. La situazione dei cristiani e degli altri gruppi religiosi in Medio Oriente, quindi, non è facile. Si stima che la popolazione di fede cristiana residente nei Paesi arabi si attesti intorno ai dieci milioni. Le comunità religiose diverse da quella musulmana vanno tutelate anche in Iraq, dove la situazione non è certamente rassicurante nemmeno dopo la destituzione di Saddam Hussein. Anzi, dalla caduta del regime ad oggi sono sorte molte nuove sette e gruppi fondamentalisti. Gli intellettuali sono stati uccisi o esiliati e sono morte 1.300.000 persone. L'iracheno Joseph Kassab, direttore esecutivo dell'Ufficio immigrazione e rifugiati in America, ha lanciato un monito molto preoccupante. Ha infatti affermato che « se le persecuzioni continuano così, nel 2025 in Iraq rimarranno solo 5 milioni di cristiani», a dispetto dei 9 milioni presenti sul territorio oggi. in questo Paese i cristiani vengono considerati filostranieri associati agli occidentali, e quindi rapiti e torturati. È una pratica comune la crocifissione e si sta diffondendo una pratica ancora più disumana. I gruppi fondamentalisti hanno preso di mira i bambini e le ragazze: ai primi viene impietosamente tagliata la testa e consegnata alle madri, mentre le seconde vengono stuprate. Esimi colleghi, potrei continuare a parlarvi dei rischi nei quali incorrono le popolazioni di fede cattolica e anche di altri culti residenti nel Laos, in Indonesia, nel Sudan, nella Nigeria, nelle Maldive, nello Yemen, nel Bhutan, in Iran, nella Corea del Nord e in tanti altri Paesi, ma penso che quanto ho finora detto sia sufficiente a farvi capire la gravità della situazione e con quale urgenza occorra affrontare il problema della libertà di culto in tutti gli angoli del mondo e la protezione delle minoranze religiose. Noi dell'Italia dei Valori chiediamo al Governo di assumere iniziative volte a contrastare la persecuzione di tutte le comunità religiose minacciate, e non solo di quelle cattoliche, come chiede la mozione presentata dal Popolo della Libertà. Siamo comunque d'accordo nel chiedere alla comunità internazionale di affrontare questo gravoso problema in maniera uniforme e procedere dunque all'armonizzazione degli interventi in materia. Non possiamo, come ultimo punto, cari colleghi, non auspicare il ricorso ad interventi da parte di organismi internazionali dei quali faccia parte anche il nostro Paese, capaci di aiutare concretamente singoli individui e comunità, la cui esistenza viene quotidianamente minacciata per motivazioni di ordine confessionale.

di questi uomini che, per non tradire la propria fede, hanno pagato con la propria vita.

È un'epidemia inarrestabile e non sarà, purtroppo, la nostra mozione a mettere fine a questo scandalo nei confronti dei cristiani. Sembra che la vita del cristiano valga il prezzo di una pallottola, perché non può essere diversamente.

è un progetto d'amore per tutti gli uomini e chi proclama il progetto cristiano è scomodo al mondo della politica.

è il fondamento della religione cristiana. L'impero romano non è finito perché doveva finire: è caduto - lo sappiamo

Il mio segretario federale da anni afferma che bisogna aiutare la gente a casa propria e che dobbiamo cercare di non farli venire a casa nostra. al di là di quello che dice il cardinale di Milano (e al riguardo apro una parentesi), che nella sua prolusione nel giorno di sant'Ambrogio

purtroppo vedo che sono i dittatori comunisti che continuano ad uccidere i cristiani in giro per il mondo. Questa è la verità. Prendete atto di queste situazioni.

il sottosuolo dell'Africa è talmente ricco e gestito da troppi dittatori che non non riusciremo a risolvere il problema africano come non riusciremo a risolvere il problema della caccia al cristiano. Il cristiano nel testimoniare la sua fede deve essere alla ricerca della verità. Questo poi è il fondamento di tutto il grande pasticcio che si vive nel mondo contro i cristiani. Il nostro Gruppo darà

sono convinta che ci sono tantissimi storici leghisti che non gli darebbero neanche il voto a partire da uno nella docimologia nella sua ricostruzione storica: storica, non ecclesiologica, non martiriologica. *(Applausi dal Gruppo PD).* E mi dispiace, sinceramente, Presidente, che un dibattito come quello che si era tenuto fino all'intervento del collega possa essere stato adesso un po' leso anche dalle nostre interperanze, ma è impossibile ascoltare ciò che non corrisponde in nessuna maniera né alla logica storica, né a quella politica, caro Sottosegretario. Pertanto, la lesione avvenuta mi rende adesso meno tenera di quanto avrei voluto essere perché in realtà, anche attraverso il suo intervento, l'Aula aveva acquisito una ricchezza di informazioni che raramente sono messe a disposizione del Paese. Purtroppo, siamo pochi noi ad ascoltare e non so quanti a leggere la sua relazione e tutti gli interventi;

mozioni. La religione appartiene all'interiorità squisita della persona, tanto che tutte le carte che hanno definito i diritti inviolabili hanno dovuto parlare della libertà religiosa. avuto senso, e non può averlo, inserire in un trattato, che si modifica a seconda della evoluzione storica, socio-politica ed economica, le radici cristiane,

stanno aumentando le persecuzioni. La Chiesa cattolica non ha problemi nel fare il suo martirologio, perché tutti i giorni dell'anno portano più o meno martiri. E sono quelli che hanno costruito quella storia per cui

Il Cristianesimo appartiene alla storia. Ci sono territori nei quali si è insediato, creando tradizione, profilo culturale e, alla fine, identità di popoli e territori. territori. Quando, però, lo si vuole attaccare in maniera antistorica, perché anche contro la dialettica storica marxiana si ricordano le crociate, di quel Cristianesimo che ha abolito la schiavitù e ha chiesto di perdonare i nemici. Questa è una norma altamente democratica perché il nemico, in democrazia, magari non lo perdoni, ma almeno non lo uccidi con le armi: tratti solo attraverso la dialettica. Il Cristianesimo ha perciò reso vero nel mondo il principio della pari dignità degli uomini, dell'uguaglianza quindi delle dinamiche relazionali. Per questo troviamo la democrazia, a prescindere dalle definizioni delle radici, lì

gli amici del nostro Governo che stanno al di là di quella che era la cortina di ferro impediscono il proselitismo. Il capo della Chiesa ortodossa in Russia, che è capo anche di una religione pubblica

ha cercato di fare di un'antropologia culturale fondata sull'umanesimo cristiano il fondamento della sua politica estera. Se con alcuni Paesi del Mediterraneo possiamo vivere con una certa serenità è anche in forza di quello. In quei Paesi c'era

per i benedettini di Tamaraset, per giustificare un eccidio, si disse che erano spie. Quindi, quando la politica interseca la religione fa valere la ragione di Stato e cancella il principio della libertà religiosa, che è una libertà inviolabile perché appartiene alla spiritualità dell'uomo: è ciò che lo rende uomo invece che altro. Allora, noi voteremo a favore di tutte le mozioni consapevolmente, perché crediamo che quando proponeva emendamenti che sembravano solo formali in realtà lei voleva impegnare questo Governo a

essere sollecitati dal Governo, che dovrebbe esercitare un po' di controllo su ciò che viene scritto, perché può incominciare ad inserirsi il principio della reciprocità: non solo in Italia, dove si chiedono le moschee, e noi le consentiamo grazie alla nostra cultura, ma anche nei Paesi in cui più proficuamente il nostro Stato esercita diritti legati agli scambi commerciali ed imprenditoriali. E poiché ciò che accade in Africa prima avviene in Italia, in Italia, il Governo viene coinvolto anche su quegli aspetti che sembrano oggi tangenziali ma non lo sono. Se c'è libertà dell'individuo e della comunità religiosa c'è libertà soprattutto dei vertici delle comunità religiose. E se a Milano ci si comporta in modo diverso da come vorremmo ci si comportasse in Africa c'è una tale, fondamentale e profonda contraddizione che non può lasciarci tranquilli. Non posso immaginare che mentre votiamo all'unanimità in questa Aula, fuori di qui si usi la religione per stabilire specializzazioni nei confronti dell'elettorato e specificità nei confronti di una cultura. Il Popolo della Libertà oggi non è tutto rappresentato in una mozione, pur importante: c'è chi non ha presentato, né sottoscritto la mozione Gasparri. È come volersi lasciare le mani libere. Per fare che? La religione riusciamo a difenderla in Asia e in Africa se difendiamo il diritto a professarla e a predicarla. Poi ognuno si comporterà secondo la propria intenzione, interiore o pubblica. Per questo motivo,

unanime e spero che ad esso seguano scelte coerenti, anche nella grande stampa, anche attraverso i *media* italiani. C'è in gioco qualcosa di più importante del solo rapporto con l'elettorato interno. Ormai la politica dei Governi su questa piccola aiuola che ci fa essere feroci riguarda l'intera Comunità. All'Europa si può chiedere, ora che ha anche la estera comune, di mettere un po' più di ambasciatori in giro per il mondo. Infatti, là dove ci sono ambasciatori che vengono da una certa cultura le relazioni diventano anche più positive. Siamo un Paese che ha al suo interno una religione che ha creato l'armonia: abbiamo bisogno che sia questo il modo di fare. Se però qui si usa la religione come un'arma, il mondo è piccolo, la televisione satellitare funziona in tutto il mondo, anche in Africa: se da qualche parte del mondo la religione divide, non si capisce poi perché in Africa non dovrebbe continuare a farlo. una nuova finestra"). Prima di passare alle votazioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione

volto a rappresentare la realtà dei quasi 5 milioni di italiani nel mondo che vivono situazioni, storie e realtà molto diverse tra loro e che esprimono anche bisogni diversi nei confronti dell'Amministrazione dello Stato; comunità italiane all'estero accomunate, però, tutte tutte tra di loro da una fondamentale funzione di promozione dell'immagine, dei prodotti, dell'economia e della cultura italiana nel mondo con incalcolabili ritorni positivi per tutta l'economia e la politica estera italiana. Il secondo obiettivo è quello di sostenere gli sforzi del Governo in un reale progetto globale di riforma della rete, dei servizi e della rappresentanza diplomatica italiana nel mondo. avvenire nel rispetto degli specifici ruoli istituzionali: il Governo ha il dovere e la responsabilità di gestione del Ministero degli affari esteri, e dunque della rete diplomatica; il Parlamento ha il dovere di rappresentare le istanze dei cittadini che lo eleggono.

È con questo spirito che abbiamo presentato la mozione. Aspettiamo dal Governo l'apertura per costruire veramente un dialogo che vada oltre la ripetuta disponibilità dell'Esecutivo a venire nelle Commissioni parlamentari di competenza ad illustrare le decisioni prese dalla dirigenza amministrativa del Ministero degli affari esteri. Da anni ormai ripetiamo un concetto basilare, secondo noi, per un piano di riforma dei servizi del Ministero degli affari esteri. Il nostro Dicastero ha una missione in più rispetto ai Ministeri degli esteri dei Paesi industrializzati. La prima è la stessa di tutti i Ministeri degli esteri, cioè promuovere il Paese nel mondo, proiettare la politica estera, l'economia, l'immagine positiva dell'Italia nel mondo. Il Ministero degli affari esteri italiano, però, ha anche la missione di dare servizi ai 5 milioni di italiani che risiedono, lavorano e vivono oltre i confini italiani. servizi che, tra l'altro, gli italiani all'estero ripagano largamente con l'incalcolabile ritorno economico che hanno rappresentato, che rappresentano e che possono ancora rappresentare in futuro per l'Italia. Ho già fornito in quest'Aula cifre ufficiali e, dunque, ne ricordo solo una: da sette Paesi europei i nostri pensionati, ex emigrati, fanno rientrare ogni anno in Italia oltre 3,3 miliardi di euro (pari a quelli derivanti da uno scudo fiscale, solo che quelli degli emigrati sono soldi puliti). degli affari esteri c'è bisogno di diplomazia; per la seconda missione c'è bisogno di servizi. Non è possibile che il Ministero degli affari esteri si autoriformi; è fin troppo evidente l'assenza di criteri oggettivi e razionali di economia ed efficienza nel piano presentato. La nostra stessa diplomazia *in loco* non è in grado di spiegare la *ratio* di tale piano e rileva pubblicamente l'assenza di economie e razionalità. Appare fin troppo evidente che si tratta di un piano principalmente ispirato ai fini degli interessi interni all'amministrazione (carriere, comodità) e non ai reali bisogni della collettività. Ripropongo qui alcuni criteri sui quali un confronto tra Governo e Parlamento non potrà che essere proficuo per il Paese: tutto, per i servizi alle comunità italiane serve meno diplomazia (non è una banalità); in secondo luogo, servono più uffici distributori di servizi, tipo agenzie, o un nuovo modello ancora più snello da costruire, da inventare, con nuove figure professionali; di assumere più personale *in loco*, con le dovute regole di gestione e di controllo necessarie a garantire la trasparenza, l'efficienza e la sicurezza dei servizi; inoltre, in Europa sviluppare i rapporti con le amministrazioni locali al fine di ottimizzare l'utilizzo delle opportunità che l'ottimo progetto presentato a Bruxelles alle Commissioni esteri di Camera e Senato dal Governo - il Sistema integrato l'esempio di accordi con amministrazioni comunali per insediare punti di servizi nelle strutture locali per gli italiani ivi residenti. È necessaria, inoltre, in una seconda fase, una riflessione politica sulla possibilità e sulle modalità per coinvolgere la fitta rete degli uffici dei patronati nel mondo. Non sono solo le comunità italiane a protestare con forza contro questo tipo di ristrutturazione. Le autorità locali hanno comunicato al Ministero degli affari esteri la loro incomprensione e il loro disappunto di fronte alla chiusura di uffici che, anche se piccoli, rappresentano sempre l'Italia. Ad esempio, il dottor Peter Müller, presidente del Governo del Saarland, che metterebbe a disposizione alcuni locali; hanno reagito le autorità di Mannheim, in Germania, il Governo cantonale di Coira, in Svizzera, e diversi altri, anche in altri continenti, ad esempio in Australia. Non posso e non voglio credere a ciò che mi viene comunicato dai rappresentanti delle nostre comunità all'estero, caro Sottosegretario. Porto qui solo due esempi: in Germania si chiuderebbe Saarbrücken per mantenere un'agenzia a Norimberga, dicono per motivi di appartenenza politica del presidente del Comites e non per la consistenza della collettività italiana; non lo credo e non credo neanche che dovremmo discutere di queste cose. Un esempio della nostra disponibilità ad affrontare gli effetti concreti di una riforma: quando lei, sottosegretario Mantica, ha trasformato il Consolato di Berna in cancelleria consolare presso l'Ambasciata di Berna, anche noi dell'opposizione comunicammo alle collettività che la scelta era coerente e che i servizi erano garantiti, e così è; ma abbiamo difficoltà a spiegare che l'allora console di Berna si è solamente trasferito all'Ambasciata di Berna: non si vedono il risparmio e la razionalità; ecco qualche esempio di difficile comprensione. Onorevole Sottosegretario, le chiediamo con spirito di collaborazione di fermare per alcuni mesi le chiusure imposte dall'amministrazione, di prendere i pochi mesi necessari alle ulteriori verifiche di funzionamento del SIFC, di dialogare con il Parlamento per progettare insieme una nuova presenza e prestazioni di servizi per gli italiani nel mondo. Le proponiamo di riaffermare il giusto primato della politica nei confronti dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri: i giusti diritti dell'amministrazione sono sacrosanti, ma non possono prevalere interessi particolari sull'interesse generale del Paese. Aspettiamo la riforma del Ministero degli affari esteri, che a mio modo di vedere non può solo essere un'autoriforma, ma deve essere l'occasione di una riflessione collettiva, perché l'immagine dell'Italia nel mondo non può essere né di destra, né di sinistra: deve essere l'immagine dell'Italia. Onorevole Sottosegretario, colgo qui l'occasione per consegnarle oltre mille firme che sono state raccolte nella nostra piccola comunità di Mannheim, quale ci chiede di ripensare le decisioni annunciate, e la informo anche che sabato scorso a Coira, nel Cantone dei Grigioni, in Svizzera, si è svolta una civile manifestazione ed oggi è in corso, sempre a Coira, una pacifica occupazione dell'agenzia consolare. Ho parlato con i nostri connazionali di Coira e mi hanno pregato di dire al Senato e al Governo che non fanno un'opposizione di principio alla chiusura di Coira, ma nella loro realtà geografica e climatica raggiungere il consolato di San Gallo, a non molti chilometri di distanza, vuol dire impegnare una giornata intera, cosa che per i nostri anziani non è una banalità. Questo è solo un esempio del bisogno di un punto di servizio e non di diplomazia. Con questo spirito di disponibilità, chiedo al Governo di accogliere la mozione così come formulata. Presidente, colleghe e colleghi, è la seconda volta che in questa legislatura l'Aula del Senato tratta una mozione sul tema degli italiani all'estero e di questo vi ringrazio e vi sono riconoscente, al di là degli esiti. Ma permettetemi di rilevare un mio disappunto sul nostro funzionamento: non capisco perché si siano contingentati i tempi di discussione delle mozioni, non vedo un sovraccarico di lavoro del Senato che lo potrebbe imporre. Su questo punto - non secondario, perché con il doppio del tempo avremmo potuto essere molto più concreti e propositivi - mi preme rilevare un passaggio dell'intervista del presidente Pisanu apparsa ieri su «la Repubblica», che cito testualmente: «D'altronde, non è casuale che l'8 aprile scorso la Commissione esteri del Senato abbia approvato all'unanimità, su mia proposta, una risoluzione sull'immigrazione e da allora attendiamo ancora che la Presidenza di Palazzo Madama la metta in discussione in Aula. Nonostante questo sia il Senato più sottoccupato della storia della Repubblica». Io condivido pienamente la riflessione del presidente Pisanu, e consentitemi anche di formulare un'ultima

una sua propria mozione, invece di aderire a quella sottoscritta dai senatori Micheloni e Bettamio, non perché il contenuto della mozione dei colleghi ci apparisse non condivisibile, ma perché riteniamo che, nell'analizzare la materia della razionalizzazione della rete degli uffici consolari all'estero, non si possa scindere lo strumento di rappresentanza, rappresentato dalla rete consolare, da tutti gli altri strumenti di rappresentanza: ovvero i Comites, i parlamentari eletti all'estero e il Consiglio generale degli italiani all'estero. Proprio su quest'ultimo organismo, il CGIE, l'Italia dei Valori ha una posizione che si differenzia da quella degli altri Gruppi parlamentari, che è stata formalizzata con un disegno di legge, a mia prima firma, che è al momento oggetto di dibattito, assieme ai progetti di legge congiunti, in Commissione affari dai colleghi Micheloni e Bettamio, nella penultima premessa, rileva che la ridefinizione delle strutture consolari deve avvenire anche tramite il contributo del CGIE, definito dai colleghi come la «massima istanza rappresentativa delle collettività italiane all'estero», e poiché come Italia dei Valori crediamo invece che il Consiglio generale (anche a seguito dell'istituzione della Circoscrizione Estero) non costituisca più il massimo strumento di rappresentanza, tanto che in un nostro disegno di legge la soppressione, con il trasferimento delle poche funzionalità ancora rimaste esclusive ai Comites, consolati e parlamentari eletti all'estero, abbiamo voluto presentare una mozione autonoma come Italia dei Valori. Detto questo, voglio precisare come vi sia, tuttavia, una grande aderenza fra le due mozioni su tutti gli altri aspetti sollevati in premessa e come vi sia anche concordia sugli impegni posti in capo al Governo. Passando all'illustrazione della nostra mozione, colleghi, non si può muovere alcuna riflessione senza aver fatto luce, *in primis*, sui tagli apportati dalle due ultime finanziarie al settore della rappresentanza all'estero. Come si legge nella mozione, infatti, è innegabile che le riduzioni delle voci del bilancio tracciate dalla legge finanziaria 2009 abbiano già significativamente penalizzato la dotazione di personale della rete diplomatica italiana, incidendo fortemente sulle condizioni operative di diversi consolati la cui attività risente principalmente di forti ritardi nell'azione amministrativa, come ad esempio nella trasmissione degli atti di stato civile ai Comuni e l'allungamento dei tempi di erogazione dei servizi. tagli vanno poi ad aggiungersi quelli apportati alla promozione della cultura, la quale non è solo il nostro biglietto da visita presso i Paesi esteri, ma rappresenta anche un forte rientro economico, grazie alla promozione del turismo verso verso l'Italia. Per far ciò è necessaria una rete relazionale di valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale, un'attribuzione a cui non possono far fronte unicamente gli Istituti italiani di cultura, anch'essi gravati dai tagli di bilancio posti in essere. Accanto a questo aspetto, sul piano delle riduzioni finanziarie, si deve poi considerare quello del 35 per cento arrecato all'insegnamento della lingua italiana all'estero, che rappresenta uno dei mezzi fondamentali per far sì che i figli degli emigrati mantengano con l'Italia un legame forte che nasce, *in primis*, dalla lingua, un legame che potrà anche agevolare un loro rientro in terra madre nel futuro. Il riordino degli uffici consolari, pertanto, non può essere discusso in un beato vuoto di contesto, ma deve essere inserito nel quadro fortemente penalizzante a livello economico che vi ho illustrato. In tale ottica, cari colleghi, credo dunque che se gli istituti di cultura italiana sono stati indeboliti, se le scuole di lingua italiana hanno subito tagli, se tutta una serie di strumenti utili per gli italiani all'estero sono stati ridotti, ecco, procedere anche con una drastica riduzione della rete consolare, chiudendo ambasciate e consolati che servono un bacino di utenza molto ampio, potrebbe essere un suicidio per l'Italia nel mondo; un ritorno all'autarchia che, oltre a ricordare drammatici periodi storici vissuti dal nostro Paese, appare totalmente anacronistico in una fase di globalizzazione nella quale l'emigrazione cresce e le relazioni estere hanno sempre più bisogno di supporto istituzionale. Siamo tuttavia consci che il progetto presentato dal Governo, che segue la manovra di razionalizzazione determinata dalla legge finanziaria 2007, deve necessariamente effettuarsi per adeguare un sistema consolare alle sfide della modernità, da una parte, e, dall'altra, alle innegabili esigenze economiche che un po' la la crisi e un po' alcune improvvide scelte del Governo hanno determinato. Tuttavia, proprio perché parliamo di razionalizzazione, ritengo che questa non possa essere attuabile con la semplice chiusura di alcune sedi, perché allora non si tratterebbe di razionalizzazione, ma di soppressione. Al contrario, la riforma dovrebbe permettere di recuperare risorse importanti per poter aprire nuove sedi di rappresentanza nei Paesi dove sussiste un nascente interesse economico per l'Italia; non solo, ma anche di adeguare la struttura consolare alla nuova forma di emigrazione che l'Italia sta vivendo: un'emigrazione che non è più quella stanziale e spinta dalla povertà, ma una emigrazione costituita dalle nuove mobilità professionali transnazionali. Per questo tipo di emigrazione, è mia opinione che servano più strutture locali, capaci di svolgere il disbrigo di piccole pratiche quotidiane e di assistere il migrante per il periodo, spesso determinato, che vive all'estero. Non a caso, nel disegno di legge che ho presentato si preferisce privilegiare i Comites, che sono diffusi sul territorio, che si occupano di reali esigenze locali e che sono direttamente elettivi, rispetto al CGIE,

dei cittadini italiani sparsi per il mondo. Pertanto, in riferimento a quanto affermato dal sottosegretario Mantica nell'audizione del 19 febbraio 2009, rispetto alle due ipotesi di riforma possibili, ossia la riduzione della rete ai soli consolati generali, oppure, al contrario, la costituzione di una rete consolare diffusa sul territorio con la soppressione dei grandi consolati, come Italia dei Valori crediamo che, di fronte ad una scelta obbligata, quella da seguire Infatti, procedere verso un accentramento delle competenze in capo a pochi consolati generali, potrebbe essere un duro colpo per le comunità di italiani residenti all'estero. In base ai dati dell'Anagrafe degli italiani all'estero, i cittadini italiani nel mondo sono più di 4 milioni, di cui 2.169.000 (il 54,1 per cento) in Europa. Su quest'ultimo dato, cari colleghi, vorrei sottolineare che, all'interno della comunità europea, dove il mercato unico favorisce l'esportazione di imprese e servizi negli altri Stati, procedere con l'annunciata chiusura di ben 13 su 18 sedi consolari non mi sembra una strategia vincente né tanto meno razionale. Sono altresì fortemente scettico sul fatto che, al momento, almeno, l'informatizzazione dei servizi consolari possa supplire alle strutture materiali e fisiche sparse in Europa. Come ho potuto appurare durante la visita dell'ottobre scorso presso il consolato di Bruxelles, nel quale è in corso la sperimentazione, la fiducia nel cosiddetto consolato digitale appare concretamente troppo ottimistica, e ci vorranno ancora anni ed investimenti perché possa davvero coprire i rapporti fra cittadini, consolati e pubblica amministrazione nazionale. Insomma cari colleghi, come afferma la mozione presentata dall'Italia dei Valori, credo che l'imprescindibile necessità di riconsiderare l'organizzazione della rappresentanza dello Stato italiano non potrà prescindere da un processo di snellimento degli organici, delle strutture e delle procedure rispetto alla situazione attuale,

di nuovi interessi strategici e commerciali non possa essere tralasciato nella ristrutturazione: penso ad esempio all'Africa, dove non possiamo chiudere ambasciate come quella dello Zambia, ma anzi dovremmo aumentare la nostra presenza sia per ciò che attiene alla cooperazione allo sviluppo, sia, come è stato sollevato anche durante l'ultimo G8, per controbilanciare i pesanti investimenti cinesi che rischiano di assumere il controllo dell'intero mercato africano. In conclusione, l'Italia dei Valori ambisce a far sì che, dal dibattito con il Parlamento, il Governo tragga quelle linee e quei principi fondamentali per approntare una riforma che consenta a chi guarda da lontano all'Italia di sentirsi orgoglioso di esserne cittadino, e di sentirsi, anche all'estero, comunque partecipe di una Nazione che sa perseguire il bene non solo di chi risiede sul suo territorio, ma anche di chi ne fa parte per diritto.

lavoratori in cassa integrazione, niente programmi produttivi. La manifestazione avrebbe dovuto essere in concomitanza con l'incontro, più volte annunciato e confermato, con il ministro Scajola. Un incontro che, soltanto nelle ultime ore, si è saputo essere stato sconvocato. Da fonti sindacali e dagli amministratori locali che saranno qui presenti domani siamo stati informati che il Governo non li riceverà. Io credo che questo sia un comportamento altamente irresponsabile, rischiosamente irresponsabile.

ultramoderni che si sono innescati in questo campo. Sottolineo che anche il cantiere navale di Palermo è in profonda fibrillazione e che domani c'è grande attesa da parte

intervenisse perché in tutte le democrazie avanzate, dove c'è un'importante produzione industriale di automobili, i Governi direttamente intervenuti e i Parlamenti hanno accompagnato, seguito e indirizzato l'azione dei Governi. È strano che in Italia i Governi sollecitino, ma sostanzialmente - come ha fatto sino adesso il Ministro delle attività produttive - svolgano una funzione notarile. Invece, abbiamo bisogno di un Governo che intervenga con intelligenza e con capacità e che faccia degli ecoincentivi

del *management* (con in testa l'amministratore delegato della FIAT) per intervenire positivamente nei confronti dello stabilimento di Termini Imerese. Signora Presidente, vi sono molte iniziative e molte proteste. Come

ogni giorno vi sono iniziative. Lunedì prossimo si preannuncia un'altra grande manifestazione proprio a Termini Imerese. Dobbiamo evitare che anche qui si arrivi a uno scontro. Bisogna prevenire, intervenire, e utilizzare le buone ragioni che oggi vi sono a favore di Termini Imerese: per il suo porto, per abbattere i costi dei trasporti e per la potenzialità di questo stabilimento collocato nel cuore del Mediterraneo.

che i parlamentari del Senato evitino poi, quando saremo in Aula, di dare un voto passivo agli ecoincentivi. Noi chiederemo che i parlamentari siciliani e i senatori meridionali, di fronte alla sfida della produzione, alzino la testa, tengano la schiena diritta e non votino a favore degli ecoincentivi se prima il piano industriale della FIAT non sarà indirizzato anche a favore del mantenimento della produzione di automobili a Termini Imerese.

Senatore Lumia, per quanto riguarda la mozione da lei presentata, tramite il suo Capogruppo, lei potrà, nella prossima riunione dei Capigruppo, ricevere una risposta relativamente a quando essa potrà essere calendarizzata. Per quanto riguarda il Governo, la Presidenza può impegnarsi a sollecitare l'intervento. Senatore Di Nardo, e chiedo l'intervento del Presidente del Senato presso il Governo e, soprattutto, presso il Ministero retto dal ministro Scajola. Domani mattina, a piazza della Repubblica, arriveranno da Castellammare di Stabia 800 operai che si

né il Ministro né un Sottosegretario domani potranno riceverli. È da quattro mesi che queste persone sono in cassa integrazione e questo comportamento da irresponsabile del Governo non fa altro che inasprire ancora di più gli animi. sono veramente molto preoccupato perché domani, insieme agli operai della Fincantieri di Castellammare, saranno presenti a Roma anche gli operai della Fincantieri degli altri cantieri italiani e non accettare di parlare con le segreterie nazionali dei sindacati di Fincantieri è veramente assurdo e inaccettabile, che potrà poi accadere domani sarà colpa solo ed esclusivamente di questo Governo. Non è possibile che per ben tre volte questi operai siano stati invitati a Roma per essere ascoltati e che, per la terza volta, domani essi torneranno nelle proprie città